Approfitto dell'arrivo del signor ministro Mastella per rammentargli un caso di cui gentilmente si è già occupato, quello del trentino Enrico Forti, detto Chicco, detenuto negli Stati Uniti - a Miami esattamente - da sette anni, per un'accusa che egli ritiene ingiusta: quella di omicidio. Entro questo mese, signor Ministro, la giustizia americana potrebbe prendere in considerazione la sua richiesta di riaprire il processo e, alla luce di nuove prove, Chicco Forti potrebbe, potrebbe, essere scagionato. Le rinnovo la preghiera rivoltale anche dai familiari, in occasione di una sua recente visita a Trento, di volersi adoperare attraverso i canali che la giustizia italiana ha anche attraverso il Ministero degli esteri per esercitare

che si ripercuote ormai con iniziative dal Parlamento europeo al Parlamento italiano da molti anni. Purtroppo c'è stato un blocco della disponibilità degli Stati Uniti dopo il caso Baraldini e io credo che il Governo dovrebbe sentirsi ancora più motivato ad intervenire in questa circostanza. Grazie, signor Presidente; grazie, signor Ministro.

I rapporti da qualche tempo non sono felicissimi per quanto riguarda lo scambio di detenuti; speriamo di arrivare ad una conclusione che auspicabilmente sia positiva per la giustizia in sé. Stiamo lavorando per questo.

Presidente. il parere potrebbe essere favorevole se vi fosse una riformulazione

riferimento non solo all'aver prestato servizio in sedi disagiate, ma anche alla valutazione dei risultati dell'attività svolta in queste sedi.

"con riferimento all'attività svolta"».

Nell'ambito della discussione generale, negli interventi del relatore e principalmente in quello del ministro Mastella, si è detto che si era pronti e disponibili a qualsiasi forma a qualsiasi forma di miglioramento

Non mi importa sapere chi è il ventriloquo, chi è il portavoce, chi è il pupazzo: quello che è pacifico è che si è modificata quella parte del testo che era stata richiesta dall'Associazione nazionale magistrati per tenere un atteggiamento di minore conflittualità nei confronti

né a rendermi in qualsiasi modo responsabile di eventuali affermazioni che possono venire dalla maggioranza: in fin dei conti questo testo è stato approvato con la collaborazione del centro‑destra, e via dicendo, anche perché, signor Presidente, lei mi deve scusare, non è che quando ho scritto l'emendamento ho ricevuto dal

ha criticato la commemorazione che ho fatto in quest'Aula, fortunatamente insieme ad altri colleghi che hanno avuto l'onore di conoscere l'avvocato Giorgio Ambrosoli.

di non dimenticare ciò che ha fatto la magistratura indipendente, ripeto indipendente,

allora

La Presidenza ovviamente

per quello che è, cioè senatore o senatrice della Repubblica. Punto e a capo. Non ci sono altre qualifiche che in questa sede possano essere date a qualsiasi senatore o senatrice. Senatore D'Ambrosio, prosegua.

Noi abbiamo difeso la nostra giovane Repubblica sia dal terrorismo nero, quando si voleva un colpo di Stato simile a quello dell'anno precedente in Grecia, sia dal terrorismo rosso. quando voleva sopraffare questa democrazia e, purtroppo, ha sequestrato e ucciso l'onorevole Moro!

(ma non da quella associata), mi sono preoccupato di proporre e far passare un emendamento molto importante e sfuggito a tanti.

di opinioni (anche con qualche eccesso che io, come avete visto, non ho mancato di riprendere, da qualsiasi parte si sia verificato), vorrei pregare i

Signor Presidente, evidentemente qualcuno nella maggioranza questa mattina ha deciso di costringere l'opposizione a cambiare quell'atteggiamento responsabile che ha assunto in questi giorni. Ma non ci riuscirà. Potrei dire tante cose sul senatore D'Ambrosio, sulla sua storia sulla sua storia di magistrato e sull'epoca non solo di Mani pulite, ma anche di quel *pool* di magistrati che usavano il mandato di cattura come elemento di costrizione a dichiarazioni e ad imputazioni. Potrei dire tante cose, come potrebbe farlo la stragrande maggioranza del Paese. Mi spiace, ma prendo atto - viva la democrazia e viva la Costituzione! che in questo momento, sul tema relativo all'ordinamento giudiziario, laddove noi lamentiamo la presenza e l'ingerenza esterna di una associazione corporativa che ha sempre tentato di condizionare l'attività del Parlamento tutte le volte in cui esso ha cercato di riformare la giustizia....

quelle dimissioni che sono state attuate giorni orsono qui, alla vigilia del nostro voto. Siamo quindi abituati a queste ingerenze esterne. È evidente che prendiamo atto - questa è la democrazia e la rispettiamo che esponenti di spicco della magistratura di quell'epoca militano in quest'Aula e ne sono espressione partecipe, prendendo parte alle procedure legislative. Non li abbiamo soltanto al di fuori del Parlamento, questi magistrati: li abbiamo anche al suo interno, perché rappresentanti di quella categoria.

ma questo è il Senato. Non siamo abituati ad assistere alla manifestazione di gesti semiosceni od osceni da parte di colleghi parlamentari. Il senatore Bettini deve chiedere scusa al Senato per il gesto che ha compiuto. Ha offeso questo ramo del Parlamento, ha offeso tutti noi. Abbia la dignità di chiedere scusa e la vicenda finisce qui. Altrimenti, signor Presidente, le chiedo di devolvere al Consiglio di Presidenza la gestione della vicenda, perché questi fatti non possono non essere stigmatizzati attraverso le doverose procedure.

che sta avvenendo in quest'Aula. Paradossalmente, mi pare che l'andamento del dibattito in questi giorni abbia dimostrato che è interesse dell'opposizione dibattere e ed è interesse della maggioranza, invece, bloccare il dibattito, in quanto è in

la democrazia del Paese, che riguarda l'ordinamento della magistratura, possa proseguire in modo ordinato e si possano confrontare gli argomenti di ciascuno di noi. Però, signor Presidente, non posso non dire pubblicamente all'Aula che quanto è accaduto poco fa non è degno di un'Assemblea

con gli argomenti opportuni che riteneva di dover portare a sostegno della sua tesi; è iniziata da parte dell'opposizione una serie di interventi volti ad interrompere il senatore D'Ambrosio. Poi è successo un fatto, signor Presidente, che non ho mai visto accadere nell'Aula del Senato della Repubblica, perché una senatrice è scesa nell'emiciclo

fermiamoci, abbiamo superato la misura. Questo non è possibile in un'Aula e in un Parlamento democratici. Queste espressioni non sono ammissibili. Credo e mi aspetto da chi le ha usate una parola di scuse nei confronti del senatore D'Ambrosio.

Quando si fa un intervento di questo tipo si ha il diritto ad una risposta. Vorrei spendere una parola sulla *bagarre*, sgradevole da tutte le parti. parti. Penso, signor Presidente, che lei non possa mettere sullo stesso piano un gesto sessista, discriminatorio, che offende la dignità di tutte le donne, con uno degli usuali

e poi tollerare in Aula un gesto patente di discriminazione sessuale. C'è una contraddizione patente in questo. Vorrei rassicurare il senatore D'Ambrosio: quest'Aula è unita nella venerazione per la memoria dei magistrati che hanno dato la vita per la difesa della legge repubblicana. Ricordo nomi come quelli di Falcone e Borsellino,

contro l'eversione di destra, e così via. Stia tranquillo, la memoria di quei magistrati appartiene a tutto il popolo italiano. Non esiste in quest'Aula un partito antimagistratura, un partito che non rispetti quella memoria. Tuttavia, non nascondiamoci dietro un dito. Esiste anche un'altra magistratura: una magistratura che ha teorizzato il diritto e perfino il dovere della politicizzazione. Esistono convegni - lei ricorderà di Magistratura democratica nei quali si teorizzava l'uso rivoluzionario del diritto e dello Stato. Ci sono libri su questo tema che lei probabilmente avrà letto

esiste una politicizzazione della magistratura che contraddistingue negativamente il nostro Paese nel contesto europeo e scuote la fiducia dei cittadini nella magistratura. Vogliamo parlarne con serietà, senza far finta che il problema non esista? Un'intera classe politica è stata spazzata via con poche sentenze di condanna, ma con tanti avvisi di garanzia, a volte con il sospetto che questi fossero accuratamente calibrati per ottenere effetti politici. Tanta gente è stata in galera e poi è stata assolta,

nell'ambito della quale la pubblica accusa è al di sopra di ogni sospetto ed esercita una funzione giudicante dentro un'unità della cultura della giurisdizione, quindi non esiste il problema di metterla sullo stesso piano della difesa, perché la difesa è sospetta e la pubblica accusa non lo è. Ebbene, questa legge, conformemente ai principi di un ordinamento accusatorio, insinua, accetta parzialmente, timidamente, quasi solo simbolicamente, l'idea che la pubblica accusa sia parte e in quanto tale debba essere sottoposta a misure di controllo e di garanzia che assicurino che non ecceda nell'uso dei poteri di parte. Questo è il tema che stiamo discutendo

perché la fiducia nella magistratura è un bene comune del Paese, allo stesso modo, però, è stato sbagliato da parte di alcuni magistrati - una minoranza, ma significativa scuotere la fiducia dei cittadini nella classe politica e nella politica, perché anche la fiducia nella politica è un bene comune del Paese. Senatore D'Ambrosio, D'Ambrosio, signor Presidente, credo che nessuno qui possa negare che questo bene è stato aggredito e scosso, e ciò è parte del problema della transizione infinita di questo Paese e della difficile ricerca di un ritorno alla normalità democratica.

Signor Presidente, ho chiesto la parola - anche se questo provvedimento viene seguito con estremacompetenza ed equilibrio dai colleghi del mio Gruppo facenti parte della Commissione giustizia, a iniziare dal senatore Caruso perché credo debba essere chiaro che il dibattito che si sta svolgendo non è pro o contro la magistratura. dibattito, alla luce dell'intervento del senatore D'Ambrosio, possa essere sulla memoria, assolutamente condivisa, di coloro che all'interno della magistratura - come ben ricordava un attimo fa il senatore Buttiglione - hanno pagato il costo della loro vita.

ma credo che nessuno, onestamente, possa disconoscere che quella riforma si inserisce in un filone di riflessioni comuni ad un'area culturale molto vasta. Basta ricordare il progetto di riforma costituzionale che prese il nome dall'onorevole Boato, approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale. Fin dall'inizio, però, la reazione dell'Associazione nazionale magistrati, e di chi se n'è fatto e se ne fa portavoce ancora oggi in Parlamento, è stata aspra e dura. Nella passata legislatura il confronto all'inizio fu aperto e reale, tant'è che nel maggio 2002, proprio su iniziativa dell'allora Guardasigilli, si arrivò ad una bozza concordata che fu poi gettata nel cestino, perché superata dalla decisione improvvisa del vertice dell'ANM di ricorrere allo sciopero, lo stesso che è stato minacciato nelle ultime ore. vorrei conoscere dai colleghi che stanno difendendo con forza alcuni passaggi molto discutibili della controriforma Mastella

Non soltanto il centro-destra, ma gran parte della cultura italiana ritiene che una moderata articolazione di carriera, basata sui concorsi, stimolerebbe la formazione professionale dei giudici e valorizzerebbe la stessa Corte di cassazione.

Non parlo poi del CSM perché uscirei fuori dal recinto, anche se la sua presenza incombe su tutto, come dimostrano e confermano le cronache delle ultime ore. Il Consiglio superiore della magistratura oggi è, al tempo stesso, legislatore con le sue circolari, giudice disciplinare con le sentenze dell'apposita sezione, amministratore con i suoi poteri di nomina e di trasferimento e, in più, rivendica con forza anche la formazione dei magistrati. È difficile, parlando da due secoli di distinzione dei poteri, trovare una così clamorosa deroga a tale principio. C'è però un profilo sul quale, con tutta onestà, il conflitto con l'Associazione nazionale magistrati è reale ed è effettivo, perlomeno da parte nostra: si tratta reale, qualche volta anche dichiarata, che la gestione politica di questo Paese avvenga nelle aule di giustizia e questo credo che nessuno, neanche il senatore D'Ambrosio, che è persona onesta, possa disconoscerlo. *(Applausi dai che il compito dei magistrati non è il controllo e l'eventuale sanzione di singoli comportamenti illeciti di singoli politici (ci mancherebbe altro!), ma il controllo e il condizionamento della politica nel suo insieme: la pretesa di bloccare qualsiasi freno posto in questa direzione, incluso il semplice divieto di iscrizione ai partiti politici. Accetto quindi la presunzione quale tutti i giudici fanno scrupolosamente il loro dovere, ma sappiamo bene che il dovere alcuni lo vedono in un modo, altri in modo diverso: alcuni cambiano concezione del dovere in base al tempo e allo spazio. La custodia cautelare, ad esempio, non viene applicata nella stessa maniera a Milano, a Roma, a Bari o a Palermo. In alcuni processi viene utilizzata la presunzione del «non poteva non sapere», in altri no. Sulle medesime carte alcuni giudici condannano, altri assolvono. Quest'alternanza fa onore all'autonomia della magistratura, ma da essa non possono dipendere i destini politici di questo Paese e i profili politici di chi riceve un mandato da parte degli elettori. In conclusione, Presidente, gli italiani leggono i giornali, vedono la televisione e constatano che ancora adesso magistrati eminenti, sovente responsabili di processi difficili e di uffici delicati, si dichiarano di sinistra, parlano come esponenti di un Gruppo politico, scrivono su «l'Unità» e su «il manifesto», tengono convegni e comizi sotto la sigla di organizzazioni politiche ben determinate. Allora, si può condividere o meno l'emendamento Palma - o come si chiamerà adesso che è stato ritirato - e si può discutere nel merito; dobbiamo però intenderci su un punto essenziale, signor il magistrato deve avere una professionalità seria e verificata e non può comportarsi come un politico di professione, per di più estremista e fazioso, a meno che coloro che in quest'Aula continuano a farsi portavoce dell'Associazione nazionale magistrati non vogliano confermare con fatti concludenti che il pericolo più grave per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura proviene dalla stessa magistratura associata. In tal caso, gli autentici difensori dell'istituzione magistratura saremo noi del centro-destra

in quest'Aula, che sta discutendo il nuovo ordinamento giudiziario, è presente un pezzo di storia, di quella storia,

Vi sono stati scontri terribili, l'Italia si è spaccata in due, si è spaccata in due, anche dentro la stessa area. Ricordo, per esempio, che nel mio campo ci si interrogava su tante cose: ditelo anche voi, però, non è possibile che abbiate soltanto incrollabili certezze. È questa l'unica cosa che in parte mi amareggia e che non riesco a seguire

ricordo come una straordinaria ma terribile esperienza, per esempio, un'assemblea che tenni all'Alfa di Arese con Caselli. Me la ricordo terribile e angosciosa ed ero lì ero lì come sindacato, come CGIL, come delegata che veniva da un'altra parte, da un'altra fabbrica. Credo che il senatore D'Ambrosio sia stato insultato non per quello che ha detto

Penso sempre che se le Brigate rosse in quell'area avessero vinto, se fossero entrate tra gli operai, non staremmo oggi qui a parlare e sarebbe successo qualcosa di inenarrabile nel Paese. È per questo e per altro ancora che sono grata a quei magistrati, anche nei momenti in cui ho avuto dissenso, ed è per questo ed altro ancora che esprimo tutta la mia solidarietà e il mio ringraziamento al senatore D'Ambrosio.

come ha visto, in questo dibattito ci siamo impegnati ad attenerci rigorosamente al testo e alla discussione. Avverto anche il dovere, in questo momento, di fare con voi in Aula tre brevi osservazioni per lo spessore e la gravità assunta dal dibattito, ma anche per i livori di fondo che emergono in una materia come questa, che ritengo costituzionalmente e istituzionalmente delicata e che richiederebbe, quindi, sobrietà e rispetto delle autonomie e dell'equilibrio dei poteri. Tre brevi osservazioni,

riconosciuto la qualità dell'impegno democratico per la crescita civile del Paese. Il dottor D'Ambrosio è stato parte importante, senatore Buttiglione, di un insieme di magistrati - Magistratura democratica e non solo - che hanno innovato in maniera positiva la giurisdizione e il diritto nel nostro Paese. Se il nostro Paese è cresciuto - e voglio dirlo qui perché li abbiamo nel nostro Parlamento e ci onorano - è perché abbiamo avuto

che in una trincea importante... *(Commenti del senatore Ferrara).* So che non vi piacciono i giudici che hanno saputo criticare i sistemi produttivi, il potere, e hanno saputo dimostrare che a volte il capitale uccide, ferisce, mutila i corpi delle lavoratrici

contro le tossicità che hanno ucciso gli operai, ma questa è la crescita democratica del Paese. Il Paese dovrebbe sentirsi garantito democraticamente perché ha avuto un controllo di legalità e di giurisdizione che è partito dalle condizioni materiali dei cittadini. È un avanzamento per tutti noi; noi non stiamo scrivendo questo disegno di legge sotto dettatura,

dei portavoce della magistratura in quanto tale. La magistratura ha una articolazione che noi abbiamo negli anni saputo conoscere: vedi i Casson, i Di Lello, i Falcone e i Borsellino, ma quanti porti delle nebbie abbiamo,

che nelle vostre parole vi è un fastidio nei confronti della magistratura in quanto tale come potere autonomo, perché è quel potere che nel nostro Paese, nella nostra Costituzione, traccia le linee del controllo di legalità e di legittimità. Allora, massima critica ad ogni sentenza, ad ogni eccesso, ad ogni incrostazione corporativa, ma rispetto della magistratura come dato fondamentale della Costituzione e della coscienza democratica del Paese.

accaduto niente di eccezionale; anzi, gli ultimi due interventi chiariscono ancor di più il fatto che dietro questa normativa che si vorrebbe approvare c'è una tifoseria politica, nel senso che vi è una convinzione giustizialista che hanno espresso i colleghi che si sono appena cimentati nel loro discorso. Come dimenticare che, per la verità, qualche critica D'Ambrosio l'ha presa

per cui l'avviso di garanzia è cosa riservata proprio alla difesa del presunto colpevole, direi presunto innocente, e dalle procure esce, prima che arrivi l'avviso all'interessato, la notizia che questo è stato interessato da un'indagine per una serie infamante di reati, che poi magari non risulteranno effettivamente veri

non è già un elemento che può creare quel risentimento popolare, non politico, da parte della gente comune, dottor D'Ambrosio?

e fosse stato eletto con un grande consenso avrebbe potuto anche dirlo. Lei, però, non può dire di essere indipendente solo perché sta qui e da qui svolge un ruolo da indipendente. Lei probabilmente è qui perché ha avuto dei meriti, non so quali, ma qualcuno l'ha nominata e il mio parere su questa legge elettorale è talmente noto che non devo spiegare perché. Essendo qui, non può allora dire di essere indipendente, politicamente parlando, e di esserlo stato anche come magistrato. Se non fosse qui, avrei rispettato questo suo autogiudizio, ma non lo posso rispettare e non la ritengo indipendente, glielo dico sinceramente. dico sinceramente. Quindi, il sospetto che non ci sia una magistratura indipendente è più di un sospetto, alle volte diventa una certezza, perché tutti abbiamo la capacità critica di analizzare.

cediamo in comodato d'uso gratuito l'Aula del Parlamento ad alcune associazioni di categoria. Vorrei chiedere ai rappresentanti di Rifondazione Comunista

dei magistrati, anzi, ne ho stima e sono amico di molti di questi e con questi critichiamo insieme l'atteggiamento politico di alcuni di loro e di alcune corporazioni. Ha detto bene la senatrice in fabbrica andavano dei vostri colleghi. Probabilmente vi chiamavate anche compagni; perché non dice anche questo, senatrice Palermi? Anch'io vado in fabbrica ad assumere responsabilmente un ruolo politico e lo fanno con me tanti altri amici, ma un magistrato è sempre tale, non può per principio declinare passioni politiche. Il giorno in cui mi dovessi incontrare, *per accidens,* con un rappresentante della giustizia e ritenere che ha un'ispirazione politica, avrei il legittimo dubbio che potrei non essere giudicato serenamente. Questo è il punto che sosteniamo. Questa è la vicenda che vogliamo difendere, che è un fatto politico di questa Aula, non un fatto politico che riguarda la corporazione, che giustamente si difende e che, grazie a collaborazioni politiche che si sono già evidenziate nel corso di questi anni chiamati Seconda Repubblica, oggi gode di appoggi, non soltanto personali, come il suo, giudice D'Ambrosio, ma anche di colleghi senatori e appartenenti a forze politiche che evidentemente qualche vantaggio da quella parte hanno avuto.

senatore Palma, dicendo che ovviamente il dibattito è stato libero. Ognuno ha espresso qui, come era necessario e doveroso, le proprie valutazioni. Devo anche dire a tutti gli intervenuti che sarà mia cura riferire al Presidente,

comprendo le ragioni che l'hanno indotta a limitare il dibattito a un senatore per Gruppo,

critica, ma se un intervento precedente avesse riguardato il merito di un emendamento e non fosse andato molto al di là, anche con considerazioni di natura personale che non sono disposto ad accettare in alcun modo, non chiederei la parola. L'avevo pregata di invitare il senatore D'Ambrosio a rivolgersi alla Presidenza e non a me.

e avrei dovuto avere la possibilità di fare mio il primo emendamento. Tutto qui, signor Presidente.

concetto si riferisce ad una valutazione inerente agli anni di attività prestati nelle funzioni che si richiedono, quindi funzioni giudicanti e requirenti con riferimento...

Dicevo, il primo attiene alla valutazione con riguardo al numero degli anni necessari ai fini del conferimento di un ufficio direttivo che si riferisce alle medesime funzioni, giudicanti o requirenti. Il secondo principio che viene inserito si riferisce all'impossibilità, per chi ha svolto funzioni semidirettive (semplifico, chi è stato procuratore aggiunto presso una procura della Repubblica), di diventare procuratore capo e, per chi è stato avvocato generale presso una procura generale della corte d'appello, di diventare procuratore generale della corte d'appello. Sotto questo profilo, non condivido le argomentazioni svolte dal collega D'Ambrosio perché, se esse possono essere valutate con favore pensando in positivo ad una possibilità di crescita professionale di un magistrato nelle varie scansioni all'interno sempre dello stesso ufficio, è altrettanto vero che, così facendo, noi precostituiamo una presenza, direi quasi a vita e per l'intera carriera, nello stesso ufficio

per poi pervenire, alla fine, a quelle di procuratore della Repubblica. Così facendo avremmo un soggetto che, nello stesso ufficio, costituirà una presenza che diventa fondamentale, insostituibile, una costante non solo giurisprudenziale ma a vario titolo. Mi chiedo: è utile, proprio in virtù delle considerazioni svolte da altri colleghi, che vi sia questa possibilità di presenza costante, questo *cursus honorum* all'interno dello stesso ufficio? A voler pensare male, penseremmo anche ad incrostazioni di potere, potere, ad una giurisprudenza che rimarrà sempre bloccata in un certo senso, ad un punto di riferimento che vedrà altri magistrati passare all'interno dello stesso ufficio ma rimarrà punto fermo per tutti gli altri. Pensiamo in particolare non tanto ai grandi, ma ai piccoli e medi uffici, ai piccoli centri di provincia in cui queste presenze diventano momenti di certezza o di dubbio sull'attività professionale del magistrato. Ecco perché, con riferimento in particolare alla seconda parte, invito i colleghi ad una riflessione: qui non si vogliono fare penalizzazioni di alcun tipo, però si vuole evitare che vi sia un dubbio su una presenza costante e su un indirizzo costante che un ufficio avrebbe attraverso questo *cursus honorum* che non è possibile assolutamente, evidentemente, bloccare. la prego di voler richiedere sia al relatore che al Governo se intendono modificare il parere e, nel caso dovessero mantenere il parere contrario, la prego di voler disporre una votazione per parti separate delle due parti dell'emendamento. Signor Presidente, innanzi tutto devo dire al Ministro che, in questa seconda fase, non mi sta aiutando molto il fatto che il Governo si rimetta all'Aula

fatti. Su questo emendamento voglio dire alcune cose molto semplici. In primo luogo, politicamente sono impegnato a difendere il testo che è uscito dalla Commissione. In

parole «funzione giudicante o requirente». Dichiaro aperta la votazione.

desideravo rappresentare ai colleghi in Aula che quanto considerato dal relatore in realtà

dai gradi più bassi fino a quello più elevato, perché, in particolare nei piccoli e medi centri, ciò costituirà veramente un problema. Qui non c'è un problema di schieramento, né possiamo scomodare la separazione delle funzioni,

punti di riferimento in positivo o negativo, che purtroppo esistono e spargono seri dubbi sulla capacità di imparzialità e di buon andamento della magistratura italiana.

euro, risultato che la disposizione determinerà. Per fare questo, signor Presidente, darò lettura dell'articolo 53 del

Orbene, per effetto di un improvvido voto dell'Assemblea, nel corso della seduta di ieri pomeriggio, quando è stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo

così dire, un padrone o una destinazione. Credo sia indispensabile, prima che l'articolo 2 venga votato nel suo complesso, che la Presidenza si faccia carico di trovare una soluzione a questa aporia.

il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 2. Mi sembra che tutta la discussione che si è svolta sull'articolo abbia trovato un punto di enfatizzazione nella proposta Manzione, talché il dibattito ha trasformato il pacifico Manzione in un grande eretico, per un questione sostanzialmente filiforme se non paradossale. E questo ci dà la misura di come non ci si possa scandalizzare, non della dettatura, ma della forte ispirazione, del grande condizionamento che l'Associazione nazionale magistrati sprigiona sui lavori di questa Assemblea. Il tramutamento delle funzioni oggetto dell'emendamento proposto dal senatore Manzione riguarda una parte secondaria dei tribunali italiani. Soltanto chi non conosce le circoscrizioni italiane può scandalizzarsi di questo modestissimo passo che è stato compiuto ieri. Oltre il 70 per cento dei tribunali italiani ha lo stesso perimetro territoriale, fra circondario e Province: questa è la verità sacrosanta. È una tempesta in un bicchiere d'acqua, è una tempesta, una enfatizzazione strumentale, è una divisione voluta, perseguita

bene, questa è la verità! Allora, se oltre il 70 per cento dei tribunali italiani ha la stessa dimensione territoriale del circondario, siamo andati ad approvare un emendamento che soltanto per 45-50 tribunali permette al magistrato di trasferirsi, anziché da Lucera a Foggia, da Foggia a Bari: questa è la grande rivoluzione che ha distrutto i sonni di una corporazione stanziale, che non si vuol muovere dal rione, questa è la sacrosanta verità!

penso sia giunto il momento di rassegnare alcune considerazioni conclusive sui rapporti tra magistratura e politica. In nel corso del dibattito tutti abbiamo assistito alle rivendicazioni di autonomia ed indipendenza della magistratura: questa è una cosa ovvia rispetto alla quale nessuno può dirsi contrario. Dobbiamo però fare una distinzione assai importante e questo lo devono sapere magistrati: l'autonomia e l'indipendenza non sono un distintivo castuale dei magistrati, ma un bene da proteggere di tutti i cittadini italiani! È l'ottica che è diversa: noi ci stiamo battendo da anni perché effettivamente l'autonomia e l'indipendenza si riverberino, attraverso l'imparzialità, nei confronti dei cittadini italiani,

che vengono - come è noto - da una carriera di funzionariato napoleonico e che hanno acquistato uno straripamento di potere nella storia del Paese che è sotto gli occhi di tutti. In secondo l'Associazione nazionale magistrati è un'associazione privata alla quale però aderisce la quasi totalità dei magistrati italiani. I pochissimi magistrati che non aderiscono sono figli senza tutela. Ve lo dico con l'esperienza che ho maturato al Consiglio superiore della magistratura: quando c'era da promuovere, o da valutare, o da sindacare l'azione di un magistrato che non appartenesse ad una corrente, ci trovavamo di fronte a un figlio di nessuno, in una terra di nessuno, se ne fregavano tutti! L'Associazione nazionale magistrati - non lo dico io, ma i costituzionalisti che si sono interessati della vita dell'Associazione e del Consiglio superiore della magistratura, non soltanto quelli in odore di centro-destra, come Guarnieri, ma anche il Pizzorusso ha parlamentarizzato e occupato il Consiglio superiore della magistratura. Il manuale Cencelli è la regola di applicazione di ogni promozione in seno al Consiglio superiore della magistratura. *(Applausi dai Gruppi

PRESIDENTE. Per favore, per stamani di incidenti ne avrei avuti anche troppi. Quindi, per cortesia, se aspettate il prossimo, fate come vi pare.

Ma una cosa è certa: basta leggere la storia del Consiglio degli ultimi venti anni per rendersi conto che quello che dico corrisponde alla verità. Non solo. I gruppi I gruppi associativi hanno i loro uffici di segretariato al Consiglio superiore divisi per correnti. Sono dei partiti. I segretari dei gruppi devono appartenere ad una stessa corrente. La divisione e la composizione dei vari uffici è rigidamente controllata dal manuale Cencelli. Cencelli sbiadisce rispetto all'applicazione certosina che se ne fa quotidianamente al Consiglio superiore della magistratura. E allora si può anche non scrivere sotto dettatura, perché tutti siamo alfabetizzati, ci mancherebbe altro, chi più chi meno, chi apparentemente e chi nella sostanza, chi con supponenza e chi con umiltà, chi con spirito di erudizione insignificante, chi studiando effettivamente, però una cosa è certa e va detta: l'ispirazione e il condizionamento che vengono dall'Associazione nazionale magistrati sono irreversibili, quotidiani, forti e questo dibattito risente di questa ipoteca. proclamare uno sciopero per il giorno20, indipendentemente dalla data e dalla collocazione temporale, per le dimensioni delle modifiche che si stanno apportando in quest'Aula, è un atto spropositato di affermazione di una primazia e di una gerarchia che non esiste nella Costituzione e che deve essere rifiutata nelle prassi. *(Applausi Da una vita mi batto perché la magistratura effettivamente acquisti, nella sostanza e nella quotidianità, i requisiti veri dell'indipendenza e dell'autonomia e li trasferisca

possano dimenticarsi che esistono pure nel nostro ordinamento norme che stabiliscono che debbono interessarsi anche di indagini a favore degli indagati. Vogliamo la eliminazione di quella contiguità che ci offende. Allora, colleghi

ma se nel frattempo il dibattito in Italia è cresciuto negli ultimi anni è perché è cresciuta la patologia dei comportamenti di certi magistrati: questa è la verità! Se certi comportamenti non avessero tracimato quotidianamente nella patologia nessuno avrebbe reclamato.

non si vogliono più schiodare da sotto casa. Basta che qualcuno di voi si legga le norme che sono state elaborate in maniera domestica dal Consiglio superiore in tema di incompatibilità per rendersi contoche un magistrato che ha figlia, nuora, fratello e avvocato nello stesso circondario non può più essere trasferito attraverso una serie di modestissime separazioni: quindi, la stanzialità è diventata il requisito quotidiano. Ecco perché si ribellano e non possono prendere il treno da Foggia a Bari e quindi hanno fatto di Manzione un eretico martire.

perché essa si realizza attraverso la magistratura e l'avvocatura.

lo spirito e l'ombra di Piero Calamandrei, nei cui confronti ormai da cinquant'anni si vanno consumando appropriazioni indebite continue. A tal proposito ricordo alla gentile senatrice Boccia che fu Calamandrei a far introdurre la componente laica nel Consiglio superiore della magistratura quando un procuratore generale dell'epoca invase un campo non di sua pertinenza, quello politico. E allora, magistrati e avvocati. E se la nostra devozione va - come ha ricordato un collega poc'anzi intervenuto - alla memoria di Falcone e Borsellino, permettete che la mia memoria vada a chi si è sacrificato in nome dell'avvocatura.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà contro l'articolo 2 perché questo articolo in realtà è stato un'occasione perduta. Non nutrivamo soverchie speranze che si potesse arrivare veramente all'attuazione del programma, non del centro-destra ma del centro-sinistra, dell'Unione, con una vera e propria separazione delle funzioni. Ma è stata un'occasione perduta proprio per il centro-sinistra, perché non è riuscito a realizzare un impianto con una sua coerenza logica e sistematica. Badate, pur non condivisibile, l'impianto originario del disegno di legge presentato dal ministro Mastella aveva una sua coerenza in una separazione molto lieve delle funzioni; aveva una coerenza anche aveva una coerenza anche il testo uscito dalla Commissione, lievemente appesantito rispetto a quello presentato dal Governo. Non ha coerenza invece il testo che sta uscendo da quest'Aula, dove c'è un salto di Regione in caso di mutamento di funzioni; ma, attenzione, se andate a svolgere funzioni civili le potete esercitare sotto casa, o comunque fuori dalla Provincia,

In realtà si è creato un vero e proprio pasticcio, a fronte di impianti che avevano una loro logica, anche se non li condividevamo perché troppo pochi rispetto ad una vera e propria distinzione delle funzioni. funzioni. Le ragioni di questo pasticcio sono evidenti. Quando il legislatore crea un testo che non ha una sua sintonia, una sua sistematicità, una sua logica coerenza dipende dal fatto che troppi fattori, troppe *lobby*

ma probabilmente l'unica vera presenza ad avere un senso, trattandosi di una riforma di struttura, era proprio quella del ministro Di Pietro, ministro delle infrastrutture.

Il centro-sinistra e il ministro Mastella hanno perso politicamente perché non hanno visto che il rilancio in realtà era un grande *bluff*. Immaginate se il ministro Di Pietro si assumeva la responsabilità di far cadere il proprio Governo: ma nel modo più assoluto! Era solo un grande *bluff*. capisco il centro-sinistra e il presidente del Consiglio Prodi. Mi sarei aspettato dal ministro Mastella, che ho sempre ritenuto un abile schermidore, la capacità di scarnificare e di abbattere un avversario abituato a ragionare e a colpire con l'accetta e non certamente con il fioretto, come è invece solito fare il Ministro. Si è arreso davanti all'accetta, peccato! Hanno perso il centro-sinistra e questo Ministro, cedendo all'Associazione nazionale magistrati, perché la trattativa non è stata svolta dal Ministro o dai Capigruppo, ma da alcuni che hanno escluso altri, subito dopo indicati nei quotidiani come nemici della categoria. Ha perso la politica del centro-sinistra, ha perso cioè quella politica di una parte del centro-sinistra che mi viene a dire: «Sono d'accordo con te, ma ho dovuto votare per coerenza di Gruppo». Ha perso la politica di alcuni dei partiti della sinistra che volevano, in assoluta buona fede, innovare, rendendosi conto delle patologie di un sistema che non verranno eliminate. Ha perso anche la politica di coloro che intendono il rapporto con la magistratura in termini di collateralismo e di contiguità, perché è una politica assolutamente miope. Quella dei magistrati è una casta non solo stanziale, ma assolutamente chiusa e questo tipo di atteggiamento si riflette nei comportamenti del loro sindacato di categoria che non esprime - ma dovrà stare attento d'ora in poi - il vero sentire della magistratura italiana. Infatti, se alle ultime elezioni del CSM ci sono state 700 schede bianche e si è registrato un minore afflusso alle urne, tutto ciò ha un significato: significa ripulsa delle correnti e degli atteggiamenti partitici e dittatoriali dell'ANM, impossibilità per il magistrato che sta fuori di essere figlio di qualcuno, come diceva poco fa il collega Buccico. Evidentemente, dunque, questa è una riforma che non può soddisfare soddisfare e che dovrà essere cambiata per renderla coerente, sistematica e per avviare quel necessario processo di eliminazione di tante patologie del sistema che noi avvertiamo, che tutti avvertiamo - che anche voi avvertite - ma che voi non volete assolutamente eliminare.

di approfondire, sul piano tecnico, i problemi che sono stati riproposti qui in Aula, nel corso di queste giornate e che si riferiscono specificamente all'articolo 2 che stiamo esaminando.

tutto comincia con la Commissione bilancio; anzi, il senatore Albonetti, relatore sul provvedimento in Commissione, chiede

al fine di verificare se si tratti di un mero aggiornamento di importi, occorrerebbe disporre degli importi tabellari attualmente in vigore».

le indennità tabellari sono ovviamente finanziate in base alla legislazione vigente, la quale finanzia anche gli aggiornamenti automatici, in quanto previsti dalla legislazione vigente,

previsto come automatico dalla legislazione vigente, il che determina che non ci sarebbe bisogno di copertura, oppure se si tratta di altra cosa. una seduta successiva, il Governo risponde a questo quesito; ovviamente mi rifaccio alle domande e alle risposte che sono state date. Naturalmente, si può sempre sostenere che si tratti di domande mal poste e di risposte non convincenti, ma debbo per forza riferire di ciò che è avvenuto, non di ciò che è giusto giusto (in questo senso, di ciò che è corretto tecnicamente; può darsi che non lo sia, perché solo chi non fa nulla non sbaglia mai). A proposito di questo punto, il Governo ‑ inteso come punto, il Governo ‑ inteso come Ministro dell'economia, lo ribadisco - risponde: «Inoltre con riferimento alle previste nuove tabelle, specifica - il Ministro dell'economia ‑ che gli importi tabellari ivi indicati costituiscono un mero aggiornamento di importi e sono quelli in vigore dal 1º gennaio 2006. Specifica al riguardo che gli stipendi dei magistrati sono assoggettati, ai sensi della legislazione vigente, ad adeguamenti triennali disposti con DPCM e che la quota aggiuntiva dell'anno 2007 costituisce un semplice acconto all'adeguamento triennale successivo». Naturalmente, vedremo che a proposito dell'acconto - qui sì - si determina un onere e che nella relazione tecnica vi è una copertura. questo per quello che riguarda la domanda - definiamola così, senatore Caruso - di ordine generale sul punto che concerne la prima, e la più importante, a mio giudizio, delle questioni tecnicamente proponibili, e cioè: questi adeguamenti stanno all'interno della legislazione vigente (trovano copertura nel bilancio a legislazione vigente) o siamo in presenza di un'innovazione legislativa che, in quanto tale, deve essere finanziata se determina un onere?

qui troviamo la risposta al quesito nella relazione tecnica, laddove si dice che l'articolo 2, al comma 11, prevede l'attribuzione del trattamento economico del magistrato ordinario in tirocinio ai vincitori del concorso per l'accesso in magistratura. L'onere che ne deriva, signor Presidente - spero di essere riuscito a farmi seguire - è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere per soli sei mesi. Su questo punto è evidente che c'è un onere, c'è innovazione legislativa, deve trovare copertura e infatti la relazione tecnica quantifica. Anche in tal caso, abbiamo ritenuto la quantificazione tecnicamente corretta, ma può darsi che abbiamo sbagliato, intendiamoci bene, però l'abbiamo valutata e, infatti, il provvedimento reca la copertura dell'onere relativo come quantificato in relazione tecnica. tecnica. In ultimo, veniamo all'argomento che è stato sollevato ieri, in particolare - sto sempre cercando di vedere se ho capito bene - dal senatore Caruso, il quale, a fronte di una

si fa riferimento ancora nella normativa, così come risulta dall'articolo, a dei commi 2 e 3 che, effettivamente, nella riformulazione dell'articolo 51 non ci sono più. Spero, senatore Caruso, se ho capito bene,

invece, nella nuova formulazione che stiamo esaminando, i commi 2 e 3 non ci sono più e c'è solo un comma unitario. Tuttavia abbiamo valutato sul piano tecnico, e c'è traccia di questa discussione nel verbale della Commissione bilancio, che, in realtà, quanto previsto sotto il profilo degli oneri dai commi 2 e 3 sia assorbito, sia cioè attratto dentro l'unico comma dell'articolo 51, dagli ultimi due periodi, in particolare da quel periodo che dice che il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva, mentre il vecchio comma 2 stabiliva che conseguono la quinta classe di anzianità i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami. L'ipotesi è cioè che le due modalità diverse determinino però in via di sostanza lo stesso effetto sotto il profilo finanziario. Naturalmente, anche questa è una tesi che può considerarsi poco fondata, ma questa è stata la valutazione. Si può sostenere il contrario - non è accaduto nella Commissione bilancio - e si può verificare. Quello che, però, signor Presidente, in ultimo debbo dire è che effettivamente, mentre tentavo di ricostruire le cose - prevedendo che mi sarebbe stato chiesto - il modo di decidere che abbiamo seguito, gli argomenti a cui abbiamo ispirato la nostra decisione, se ce ne fosse il tempo come minimo bisognerebbe sostenere che c'è un problema, senza che ci si determinino maggiori oneri, di coordinamento della norma. Quindi, o in sede di coordinamento oppure attraverso una breve sospensione che possiamo fare nell'intervallo, non so quando,

vigente del riferimento ai commi 2 e 3 che nella legislazione come modificata non ci sarebbero più. Secondo me, dal punto di vista finanziario non cambia nulla, ma dal punto di vista della corretta interpretazione della norma, effettivamente il problema ci sarebbe.

l'articolo 2 debba essere accantonato in modo che nell'intervallo, nella sospensione dei lavori, possa essere valutato in sede di Commissione e nel frattempo si potrebbe procedere con l'articolo 3 e successivi in attesa del pronunciamento sull'articolo 2 che è *sub iudice* della Commissione bilancio. Colleghi, credo sia necessario comunicare all'Assemblea che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ribadisce all'unanimità che come termine ultimo, domani alle ore 11,30, inizieranno le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge n. 1447.

Signor Presidente, confermo che presso la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità si è raggiunta questa intesa, che peraltro costituiva il fulcro dei nostri ragionamenti, avvenuti nelle precedenti riunioni Vi è stato sempre l'impegno dell'opposizione a garantire che l'Assemblea esitasse un testo sull'ordinamento giudiziario entro questa settimana. Questo impegno viene confermato e ribadito anche in Aula. Quindi, facciamo proprie le dichiarazioni del Presidente che, a nome di tutti i Gruppi, ha espresso il deliberato della Conferenza dei Capigruppo. Ove, entro la giornata di domani e l'orario indicato dal Presidente, non si fosse pervenuti al voto finale, da quel momento scatteranno le procedure di armonizzazione dei tempi per fare in modo che l'Assemblea, entro la metà della giornata di domani, dia il voto finalmente complessivo su tutti gli articoli.

diciamo che questo articolo 3 non è sicuramente fra quelli che comportano una forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione, perché in qualche modo l'impianto originario della riforma è stato fatto salvo. Ci sono però due questioni fondamentali che sono state modificate, per le quali vorrei avere una delucidazione, possibilmente dal ministro Mastella. la seguente: viene istituita questa figura del segretario generale della quale francamente non si vede la necessità, soprattutto in un momento in cui la politica è accusata di aumentare esponenzialmente il numero delle cariche, le spese e quant'altro. Andiamo a a prevedere una figura che non era prevista nel disegno di legge originario e che va ad aumentare il numero dei burocrati dello Stato. È vero che si dice che il segretario generale non deve avere alcuna ma è altrettanto vero che un segretario generale di una scuola avrà sicuramente diritto ad una segretaria, ad un ufficio e all'auto blu, perché ovviamente non si può negare a nessuno, e quindi sicuramente le spese aumenteranno.

*benefit* ai quali evidentemente non può rinunciare, pena la sua non funzionalità, e che invece non sono previsti. La seconda questione, quella molto più importante, è la variazione della destinazione delle sedi della scuola. Anche

sia importante che il magistrato faccia parte del contesto territoriale nel quale si trova ad operare. In questo senso avevamo individuato tre sedi sparse e diffuse sul territorio nazionale, in modo che ci fossero delle scuole a cui la magistratura, gli uditori e tutto coloro i quali volessero utilizzare questa scuola, che doveva essere un organo aperto, potessero far riferimento. Bene, questa dizione è scomparsa. Si parla semplicemente di tre sedi, che potrebbero essere, a questo punto, tutte e tre in Sicilia, in Trentino o in Friuli, alterando completamente la *ratio* della norma. Vorrei capire se si tratta di una svista, ma non credo, perché ho già avanzato questa osservazione in Commissione, ma mi è stata data una risposta non esaustiva. Vorrei che su questo punto invece ci fosse un chiarimento, che mi pare sia molto importante. Tra l'altro, il mio emendamento ribadisce una questione - è un po' strano che lo dica un federalista come me, ma credo sia una questione razionale la sede principale deve essere evidentemente nel contesto dell'Italia centrale, anche per una semplice questione di baricentro geografico, mentre invece anche su questo punto la norma, così com'è scritta e novellata in questo testo, non dice nulla.

Posto che all'articolo 5, con posizioni e funzioni del Comitato direttivo, è scritto che «il Comitato direttivo adotta lo Statuto», mi sembra di tutta evidenza, signor relatore, che adottandolo egli abbia e debba avere anche competenza a modificarlo, perché altrimenti in caso di errore, chi lo modificherà lo statuto se non chi l'ha scritto? della giustizia*. Sui rilievi che ha formulato il senatore Castelli debbo dire che l'indicazione di un segretario ha una funzione di natura organizzativa,

Presidente, signor Ministro, colleghi, stiamo trattando un emendamento a favore del Ministro. Il ministro Mastella in questa occasione ci ha particolarmente meravigliati perché è il primo Ministro a rinunciare a una fetta di potere (non intendo definirla tale), ma a una posizione del proprio Dicastero nell'ambito della scuola. Vi erano posizioni paritarie: Consiglio superiore della magistratura, Ministro, con il concorso del mondo dell'avvocatura e dell'università. Inopinatamente il Ministro rinuncia ad una propria posizione nella possibilità di designare e nominare questi componenti in favore del Consiglio superiore della magistratura. Allora, a poco vale la sua giustificazione che comunque il Consiglio superiore della magistratura è fatto da alcuni componenti eletti da magistrati e altri dal Parlamento. Si tratta di un organo che poi nella sua complessità si caratterizza come tale. Devo dire che ci ha meravigliato, che continua a stupirci - come suol dirsi con una banalità - con effetti speciali. Aggiungo che mi sembra strana, onestamente, questa disparità e questo depotenziamento del ruolo del Ministero all'interno di una Scuola di formazione che nessuno vuole sbilanciata a favore dell'Esecutivo, ma che deve vedere organismi di rango costituzionale, con compiti diversi, egualmente rappresentati.

non tutte le norme che sono state fatte devono avere spiegazioni dietrologiche. Questa modifica, come si ricorderà, l'ho proposta io

designati dal Ministro e sei dal Consiglio superiore della magistratura, d'intesa tra loro; quindi vi lascio immaginare cosa sarebbe accaduto. Allora si è tolta la formula «d'intesa», per cui le nomine del Ministro avverranno in maniera autonoma. A quel punto, è anche giusto che ci sia una certa riduzione delle sue nomine, anche perché, come ricordava lo stesso del Consiglio superiore della magistratura fa parte pure una componente laica della quale abbiamo autorevoli rappresentanti anche in questa sede. Naturalmente, questo non deve far trasparire una voglia di lottizzazione che purtroppo, come diceva il senatore Buccico, non è infrequente in quel campo ma, diciamoci la verità, non è infrequente neanche nel campo di noi politici; quindi, prima di gettare la croce sugli altri vediamo anche come ci muoviamo noi. Dunque, siccome anche nella che deve essere ovviamente imparziale, non politicizzata, si esprimono indirizzi culturali diversi, è giusto che in questa scuola, molto importante perché provvede alla formazione della magistratura,

che ha insospettito il collega Centaro, ma quella più significativa, a mio avviso, è l'eliminazione del criterio dell'intesa, che avrebbe spinto ad una inevitabilmente deteriore contrattazione tra magistratura e Ministro sulla funzione di questo organo.

il rilevante esempio di onestà intellettuale e di libertà fornito dai colleghi della Commissione giustizia del Senato e e dai colleghi di maggioranza presenti nella Commissione stessa. Infatti, l'approvazione di un emendamento in quella sede ha consentito, per la prima volta nella nostra storia, che un apparato destinato ad occuparsi di giustizia, quale sarà la Scuola superiore della magistratura, non risulti autoreferenziale alla magistratura stessa, ma possa aprirsi a un pluralismo di esperienza, e in particolare di esperienza amministrativa.

Il segretario generale della Scuola superiore della magistratura, quindi il massimo organismo organizzativo della stessa, potrà essere un magistrato o, in alternativa, un dirigente generale dello Stato, cioè un soggetto che, istituzionalmente, si occupa delle mansioni tipiche di un segretario generale.

per quanto concerne la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3, comma 10, il Ministero fa presente la neutralità finanziaria della previsione che, nell'ipotesi in cui si intenda nominare un dirigente di prima fascia, può ritenersi assicurata a condizione che la designazione ricada su un dirigente di prima fascia attualmente in servizio. In tal caso, suggerisce

«Il Presidente Morando evidenzia che la previsione della possibile elezione di dirigenti di prima fascia appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi, per cui non appare convincente la posizione espressa dal Governo, risultando invece necessaria una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». Così sarà poi redatto il parere e così il presidente Morando calerà la mannaia dell'articolo 81 su questa apertura secolare all'interno di un sistema che era sedimentato e che tale rischia di rimanere. Ieri sera ho ascoltato il presidente Morando quando, al termine della seduta, ha detto che non interverrà mai in Aula per dare spiegazioni e, possa condividerlo o no, senz'altro lo capisco.

di volta in volta nei resoconti dei lavori della Commissione bilancio. Ora, il presidente Morando vorrà riconoscere che in questo resoconto della Commissione bilancio che ho letto non vi è alcuna motivazione del suo assunto: «La previsione della possibile elezione di dirigenti di prima fascia appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi». Ho detto prima che sono irriducibile e i colleghi si dovranno abituare o scusarmi.

avevano detto loro che (mi correggerà, poi, il senatore Albonetti se riferisco in maniera non appropriata quello che lui mi ha detto e comunque quello che io ho capito) capito) se viene nominato un direttore generale di prima fascia, inevitabilmente si determina una scopertura in una posizione - quella occupata da quel dirigente che determina la necessità di essere ricoperta e quindi la necessità della nuova spesa; su questo punto avrebbe senz'altro ragione il senatore Morando. Presidente, lei per primo mi scuserà per la irriducibilità, ma sono andato a cercare il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non è tra le mie passioni, ma riguarda le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Agli articoli 19, 23-*bis* e 23 c'è scritto l'esatto contrario di quanto è stato suggerito ai commissari e al presidente della Commissione bilancio. bilancio. All'articolo 19, comma 10, si dice: « dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione» E ancora: «Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministro degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra i livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti». L'articolo 23 recita: «È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili in base all'articolo 30».

a domanda possono essere collocati in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di attività presso soggetti, organismi» e così via. Questa, signor Presidente, è la prova provata che esistono - ma è cosa che sapeva, per la verità, chiunque dirigenti di quelli che abbiamo considerato "a disposizione", come dice, cioè che possono essere utilizzati. Ma è una ovvietà, signor Presidente, il sistema ce lo insegna. Devo allora chiedere al presidente presidente Morando e alla Commissione bilancio, magari utilizzando la pausa dei lavori per uno spazio di lavoro, di riconsiderare il parere su quel testo votato dalla Commissione giustizia, al Ministro di ritirare questo emendamento. Mi riservo per il futuro, quando avremmo più tempo, di fare qualche riflessione sul funzionamento del nostro Senato, in relazione al quale sono già intervenuto per altro argomento questa mattina.

Però non posso ritirare il mio emendamento fino a quando la Commissione non formuli un articolato che trovi questa soluzione. PRESIDENTE. Presidente Morando, Presidente, ricominciamo da capo.

però non funziona così di solito. Dico solo questo, poi vediamo tutto quello che si può fare. Vorrei dare una spiegazione ai colleghi, perché apparentemente gli argomenti del senatore Caruso sembrano convincenti. Signor Presidente, siamo alle solite. C'è una norma che prevede che esista un'attività di direzione svolta da qualcuno che è negli organici di una amministrazione, in questo caso gli organici della Giustizia. Naturalmente, in quella ipotesi, questa figura e l'attività di questa figura sono coperte dal bilancio a legislazione vigente. Il Parlamento, in piena legittimità, esamina l'ipotesi di attribuire questa funzione di direzione ad una figura - un direttore generale

che, se prendo un direttore generale, che attualmente sta dirigendo un dipartimento della pubblica

se in quel posto metto un direttore generale che sta dirigendo un dipartimento della pubblica amministrazione, in quel dipartimento non c'è più il direttore generale. Siccome devo presumere che i direttori generali a qualcosa servano (anche se nella realtà spesso ho qualche dubbio, ma non sono legittimato ad averlo quando svolgo

dell'amministrazione non dovrebbero variare le previsioni di bilancio, perché comunque è un funzionario che già esiste; in realtà, non è così perché si scopre un posto e, quindi, si presume che quel posto debba essere poi coperto, per cui bisognerà assumere un nuovo funzionario con onere a carico dello Stato.

nella formulazione in cui è stato proposto l'emendamento del Governo, che taglia la testa al toro con tutta la bestia. Credo che il Governo possa sottoporre una formulazione che possa far vivere le intenzioni della Commissione senza ricadere negli strali della Commissione bilancio. CASTELLI *(LNP)*. Quindi, in ogni caso, noi riceveremo un parere dalla Commissione bilancio alla ripresa dei lavori dell'Aula.

l'articolo 4 si riferisce alle problematiche attinenti al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, di nuova istituzione, istituto istituto omologo al Consiglio giudiziario presso la corte d'appello, riconoscendo alla Corte di cassazione una dignità ed un valore diversi rispetto alle attività di merito, come d'altra parte è più che logico pensare, e quindi anche ai fini della valutazione, considerata la diversità tra la valutazione di funzioni di merito e la valutazione di funzioni di legittimità che necessariamente da ciò deriva. Il punto centrale su cui si è imperniato il confronto tra Commissione e Aula riguarda la presenza degli avvocati

la natura e il tipo di deliberazioni alle quali possono partecipare. Si è cominciato con difficoltà e, in un primo tempo, lo stesso Comitato aveva espunto la partecipazione al Consiglio direttivo della Corte di cassazione del presidente del Consiglio nazionale forense. D'altra parte, nel momento in cui vediamo il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la stessa Corte esserne componenti di diritto, in sintonia con quanto si verifica nei Consigli giudiziari presso le corti d'appello, dove sono membri di diritto il presidente della corte d'appello e il procuratore generale della Cassazione, logica vuole che in rappresentanza dell'avvocatura sieda il massimo massimo vertice, l'esponente apicale della categoria, vale a dire il presidente del Consiglio nazionale forense. sintonia e sistematicità, non può che avvenire presso i Consigli giudiziari, dove logica vuole che la rappresentanza dell'avvocatura veda la presenza necessaria del presidente del Consiglio dell'ordine del luogo. Tuttavia questa logica sembra essere scomparsa in virtù delle solite pressioni dell'Associazione nazionale magistrati. Infatti, nel momento in cui si arriva alla possibilità che il presidente del Consiglio nazionale forense sia componente del Consiglio direttivo della Corte

Corte. Tutto ciò avviene perché il componente di diritto, per logica sistematica del nostro ordinamento, non può che partecipare a tutte le delibere e a tutte le decisioni dell'organismo di cui è componente di diritto. Questo avrebbe comportato, in tutta evidenza, che il presidente del Consiglio nazionale forense avrebbe potuto partecipare anche alla valutazione dei magistrati. Apriti cielo! Ho sempre sostenuto che i migliori giudici dei magistrati siano gli avvocati. Non ho assolutamente paura di essere valutato da un consesso forense. forense. Mi riferisco infatti ad una categoria intesa sempre nell'accezione migliore, e certamente vedo in coloro che ne sono rappresentanti una rappresentanza responsabile e non messa lì per consumare vendette o per badare alla piccola bottega; anzi, per migliorare un sistema che alla fine va a favore di tutti, non solo dei magistrati e degli avvocati, ma soprattutto dei cittadini, veri destinatari del servizio giustizia. Allora non si comprende, se non a fronte di una chiusura corporativa e di casta, la possibilità che due componenti della classe forense, quindi non un numero in grado di spostare gli equilibri in caso di difformità di vedute e in caso di votazione, ma soltanto due, possano partecipare a queste deliberazioni.

sia stata messa da parte, in nome di una chiusura corporativa miope, che vede nell'esclusivo foro domestico la possibilità di valutare i colleghi. Le valutazioni dei colleghi da parte del Consiglio giudiziario sono tutte infarcite di superlativi assoluti: appena vi è un superlativo relativo, si comincia a pensare che, forse, qualcosa non funziona. Da qui le ragioni di una riforma dell'ordinamento giudiziario di cui anche questo testo, comunque, non riuscirà ad eliminare

importa la circostanza che il Consiglio dell'ordine possa comunque segnalare fatti che hanno attinenza con deviazioni nell'attività del magistrato, con patologie del sistema. Poco importa, ugualmente, che possa produrre una relazione al riguardo, o comunque una relazione sulla figura del magistrato, perché poi, alla fine, ci sarà sempre la chiusura domestica e la giustizia domestica che valuteranno tutto ciò. È fin troppo evidente che la presenza del presidente del Consiglio dell'ordine e del presidente del Consiglio nazionale forense

proveniente dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e quella proveniente dal Consiglio nazionale forense, con riferimento all'attività di quel magistrato. Non si è voluti arrivare a ciò e non lo si è fatto anche con una certa miopia. Infatti, nel momento in cui si elencano i titolari di tre funzioni (il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense) tra i componenti e li si individua nominativamente, con riferimento all'ufficio di cui sono titolari, è chiaro che, se anche non vi è la definizione esplicita che si tratta di membri di diritto, tali sono, in realtà, a tutti gli effetti, perchè diversamente

caso una delegittimazione e un'offesa nei confronti della classe forense, che ha dato e continua a dare un validissimo contributo all'amministrazione della giustizia e che ha pagato, anche con il sangue, la propria attività a difesa della legalità e delle istituzioni.

Abbiamo esaminato, all'articolo 1, le novità, per la verità pochissime (quasi inesistenti), sulla carriera dei magistrati. Sull'articolo 2 la delusione è stata totale: anche il più timido accenno di separazione delle funzioni è stato distrutto dal cosiddetto emendamento Brutti. L'articolo 3 ha riguardato la Scuola superiore (e sentiremo cosa ne pensa la Commissione bilancio): il tentativo di renderla una cosa seria è miseramente fallito, perché si trattava di mettere finalmente il bavaglio alle presunte scuole che si muovono da tante parti per formare i magistrati. Tratteremo seriamente in finanziaria questa norma antispreco: l'attuale maggioranza vuole sprecare tutti i soldi a favore dei propri amici (e anche la Scuola superiore è fatta di sprechi per i propri amici). L'articolo 4, però, comporta un problema di ordine costituzionale molto serio:

i quali non esiste neanche la distinzione delle funzioni. Questa è una legge contro gli avvocati; è una legge di insulto agli avvocati come categoria; è una legge che non riconosce la qualifica di diritto a presidente del Consiglio nazionale forense in materia di giudizi per l'esame davanti alla Corte di cassazione.

ritengo però che non sarà approvato neanche quell'emendamento, avendo già detto il relatore che è contrario, e il Governo, addirittura, ha detto che si dimetterà se sarà approvato. Potete immaginare voi che fine farà quell'emendamento. Voteremo l'emendamento Manzione, chiedo ai colleghi di votare i due emendamenti presentati da me; voteremo tutti gli emendamenti che tendono a stabilire un minimo di dignitosa presenza dell'avvocatura nel contesto della giustizia italiana. Se così non sarà, ne prenderemo atto, ma, ripeto, non vi meravigliate che poi la gente vi giudica male.

le resistenze che sembrano esservi nella maggioranza all'allargamento dei Consigli giudiziari anche agli avvocati, quasi che nel Consiglio superiore questa esperienza già non vi sia, quasi che nell'organo di autogoverno della magistratura, che per l'appunto è deputato tra l'altro alle valutazioni dei magistrati, non siano presenti personaggi esterni alla categoria dei magistrati e, segnatamente, avvocati e professori universitari in materie giuridiche nominati dal Parlamento. E che prima questa previsione non vi fosse era la diretta conseguenza del fatto che i Consigli giudiziari non avevano i compiti che attualmente invece hanno. Quei compiti che mano a mano sono stati decentrati dal Consiglio superiore per rendere in linea di massima più efficace l'azione dell'apparato di autogoverno. Si dice che gli avvocati non possono essere presenti nel Consiglio giudiziario perché in qualche modo potrebbero, essere essere momento di pressione indebita nei confronti dei magistrati. Ritengo personalmente che non sia così, ritengo che questa sia una scusa, sia un alibi. La realtà vera è che gli avvocati non possono essere presenti nei Consigli giudiziari perché i magistrati, attraverso i Consigli giudiziari, intendono restringere la loro categoria, vogliono fare e disfare della vita dei magistrati senza che vi sia una voce esterna. Davvero voi pensate che sia del tutto inutile la presenza degli avvocati all'interno dei Consigli giudiziari, che davvero sia inutile una responsabile voce di chi quotidianamente è a contatto con i magistrati e quotidianamente è in grado di valutare il loro equilibrio, la loro professionalità, la loro capacità? La chiusura agli avvocati dei Consigli giudiziari è, quindi, conseguentemente un mantenere un privilegio, è un discorso di casta. E la cosa singolare è che, quando taluni comparti associativi erano assai lontani dalla gestione dell'organo di autogoverno, bene, quei comparti associativi, e faccio riferimento a Magistratura Democratica, richiedevano a gran voce l'allargamento dei Consigli giudiziari a voci esterne, ivi compresi gli avvocati. Credo sia invece fondamentale la presenza degli avvocati, anche perché oggi vi è stata una denuncia in quest'Aula. Una denuncia di notevolissima gravità, signor Presidente. Il senatore D'Ambrosio

è. Trovo davvero grave che un'accusa così pesante nei confronti della magistratura provenga da chi ritiene di essere uno

al di là delle concezioni sulla democrazia, posso pur dire che se la magistratura indipendente è quella che, secondo la senatrice Palermi, frequenta le riunioni sindacali e quant'altro, in verità

tutta. Sempre nel corso di quell'intervento il senatore D'Ambrosio ha affermato che, grazie a quella magistratura indipendente, che va per fabbriche, molti di voi

molti senatori hanno il privilegio di sedere in quest'Aula. Immagino che il discorso del senatore D'Ambrosio fosse nel senso che quella magistratura indipendente, diversa dall'altra negativa,

Mi permetto così sommessamente di dire, signor Presidente, ma senza che questo possa suonare polemica, che forse la magistratura, quella seria, quella vera, ha lottato in questo Paese contro i fenomeni criminali, che sicuramente i signori che siedono in Aula siedono in Aula lo fanno in ragione del consenso elettorale e che probabilmente qualcuno siede in Aula solo perché ha fatto parte di quella magistratura, definita indipendente. e LNP).* Sono profondamente laico ed, essendo tale, nutro la più grande tolleranza nei confronti e nei riguardi di qualsiasi credenza

Allora, cerchiamo di essere chiari una volta per tutte: siamo al Senato della Repubblica. Ciascuno di noi porta con sé il frutto delle proprie esperienze lavorative, sociali, culturali e civili, ma l'avere o non avere fatto determinate cose non è qua dentro né punto di merito né punto di demerito. E molto poco importa se qualcuno ha sostenuto o meno certi processi. In verità, se uno volesse fare un'analisi generale, come ho già detto qualche giorno fa, scoprirebbe

quella alla quale mi onoro tuttora di appartenere, ha fatto per questo Paese: i morti che ci sono stati, i grandi sacrifici. Però mi permetto di dire, anche con riferimento a quel momento di felicità che il ritiro di un mio emendamento le ha dato, che quando c'era da contrastare

quando c'era da contrastare la criminalità organizzata io c'ero, quando si trattava di lasciare la comoda sedia romana o milanese per andare in Calabria io c'ero. Qualcun altro, invece, no.

Signor Presidente, vorrei esprimere in breve la posizione del mio Gruppo, che è favorevole al mantenimento del testo della Commissione

un dibattito acceso ed interessante, ma non sempre, per la verità, volto a questioni che avessero effettiva rilevanza svolto con un'intensità sicuramente maggiore di quella che la rilevanza oggettiva delle questioni avrebbe suggerito o richiesto. Abbiamo visto nascere e manifestarsi una sorta di ipersensibilità su temi di sicuro importantissimi, come l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma che pure comporterebbero valutazioni in ogni caso pacate, perché non è giusto vedere una qualunque decisione normativa

sono volte al più efficace svolgimento della funzione nel suo complesso, svincolando quindi il ragionamento legislativo dalla tentazione di prendere le armi all'attacco o a difesa di questo o di quell'altro. Guardando adesso alla questione dell'articolo 4, penso che non sia in alcun modo possibile avere dei dubbi è giusto e utile che gli avvocati abbiano un ruolo nella valutazione dell'attività dei magistrati? Non credo che ciò si possa negare, né penso che il fatto che gli avvocati abbiano un ruolo in tale valutazione possa in alcun modo costituire lesione del principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La questione però, tradotta nei termini dell'articolo 4, è se è utile e opportuno che gli avvocati svolgano tale ruolo partecipando al Consiglio giudiziario, che, come ovvio, è altra e diversa questione.

Non è detto che la scelta migliore e la via più utile sia quella di andare al condizionamento dall'interno, piuttosto che non avere una scelta in una chiave di diversità. Penso che sia questo il punto di valutazione dell'operato della Commissione, che fa una scelta, opinabile non c'è dubbio, ma sicuramente non riferibile allo scontro epocale che qui si può vuole prefigurare. La scelta della Commissione, che non vuole affatto negare il ruolo degli avvocati, è quella di ipotizzare se la valutazione da parte del ceto forense dell'attività di magistrati e del magistrato, giusto e utile come dicevo, debba seguire un diverso percorso valutativo. Un diverso percorso valutativo che non si svolge all'interno di organi di concertazione è la premessa di una più efficace valutazione della bontà del servizio nello svolgimento della funzione, dell'efficacia del servizio erogato. La scelta della Commissione non è affatto da intendere come un insulto agli avvocati, come diceva prima il collega D'Onofrio. Questo non è sicuramente vero; è piuttosto una richiesta agli avvocati di svolgere fino in fondo nei modi più efficaci e non in modi concertativi

A questo punto, considerata la dimensione dell'articolo 4 e il tempo che ci resta, chiuderei la discussione sull'articolo e rinvierei la votazione degli emendamenti alla ripresa, dopo l'esame dell'articolo 2 e 3 per l'emendamento che ci rimane. Passerei quindi all'articolo 5, sul quale vi è una proposta di stralcio da parte della Commissione. Ovviamente, proponendo lo stralcio, credo esprima parere favorevole.

di fare lo stralcio dell'articolo 5 in maniera che oggi pomeriggio si potesse passare alla votazione, secondo l'ordine che deciderà la Presidenza, degli emendamenti accantonati e dell'articolo 4. Se questa è la proposta, Presidente, mi pare ragionevole, e probabilmente si è creato un equivoco con il collega D'Onofrio, altrimenti anch'io condivido la sua conseguente soluzione di continuare nella

il voto sull'articolo 2 dopo il necessario approfondimento in Commissione bilancio sul problema sollevato dal senatore Caruso.

il medesimo quesito da risolvere in Commissione bilancio rispetto all'emendamento 3.800 su cui il Ministro si è impegnato a trovare una soluzione alternativa e, in seguito, si voterà l'articolo 3.

di sospendere la seduta per dare modo al collega Morando di convocare la Commissione bilancio e dare i pareri che ci sono necessari per poter proseguire.

oltre che per definire la questione che è stata a lungo dibattuta ieri in quest'Aula (questione assai importante, signor Presidente, per quanto riguarda la possibilità dei senatori di organizzare il proprio lavoro soprattutto in fase emendativa), anche per definire esattamente l'interpretazione dell'articolo 76 sul quale io sollevai un quesito al Presidente del Senato. L'articolo 76 riguarda la temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati, che è materia assai simile a quella discussa ieri in ordine agli emendamenti. Si tratta di disegni di legge e non di emendamenti ma, appunto, in materia assai simile. Poiché sul mio quesito il Presidente del Senato disse che avrebbe convocato la Giunta per il Regolamento per dare una interpretazione assolutamente coerente con quella che poteva essere una prassi chiara per il Senato e quindi anche per i senatori, vorrei pregarla, signor Presidente, di sollecitare il Presidente affinché convochi la Giunta per il Regolamento su queste questioni. Quello che ieri abbiamo discusso in Aula è un argomento di grandissima rilevanza perché il fatto che possa essere discusso un emendamento il cui contenuto, sostanzialmente, è stato bocciato precedentemente dall'Aula, lei comprende come possa sicuramente stravolgere le nostre abitudini di lavoro in quest'Aula. Poiché noi siamo assolutamente del parere che più chiare sono le regole e meglio lavoriamo, volevo pregarla, appunto,

i commi da 1 a 7 dell'articolo 5, ad eccezione della lettera *b)* del comma 2, costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Modifiche al decreto-legislativo n. 240 del 25 in materia di competenze dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari nonché di decentramento dell'organizzazione giudiziaria» commi da 5 a 18 e da 20 a 25, il comma 26, lettera *b)*, ed il comma 27, nonché i commi da 36 a 45 e da 49 a 51, oltre ai commi 53 e 54 dell'articolo 6, costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione giudiziaria» il comma 1 ed i commi da 28 a 32 dell'articolo 6 costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Disposizioni in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura»

«Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare norme di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare ed in materia di transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria»